in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Sottosegretario di Stato e professore universitario, è scomparso a Roma il 30 aprile scorso a 79 anni. Nato a Scafati, in provincia di Salerno, il 17 ottobre 1936, si sentì sempre profondamente legato alle istituzioni e in particolare al Senato. La sua carriera parlamentare quasi trentennale, infatti, inizia e termina in questa Camera. In Senato entrò come subentrante agli inizi dell'VIII legislatura, iscritto al Gruppo parlamentare Democratico Cristiano. Nella IX legislatura fu rieletto senatore nelle fila della DC per il collegio Foligno-Spoleto. Pur non essendo umbro d'origine, riuscì a creare con l'Umbria e il suo elettorato un legame molto forte nel corso degli anni. Anche questa circostanza era la misura di come Saporito intendesse l'attività politica: non un fatto autoreferenziale, bensì un servizio responsabile nei confronti della società e soprattutto dei ceti più deboli, come ebbe a dire in un dibattito in Senato. Il legame stretto che fu in grado di creare con la terra e le popolazioni umbre gli valse la rielezione al Senato, sempre nella stessa circoscrizione, sia nella X che nella XI legislatura. Durante la X legislatura gli fu affidato il primo incarico di Governo quale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel primo Governo Goria e poi nel Governo De Mita fino al 1989. Fu quindi nominato nello stesso Esecutivo Sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica, incarico che gli venne rinnovato nei Governi Andreotti sesto e settimo. Già componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione affari costituzionali nella XI legislatura, assunse altresì la carica di Vice Presidente del Gruppo della DC e fu nominato membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Pur non rieletto nelle due successive legislature, non smise mai di occuparsi di politica e della cittadinanza, anche nella sua veste di Presidente dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati dal 1981 al 2010. Negli anni Novanta si dedicò con maggior vigore all'associazionismo e all'attività politica locale, essendo anche assessore alla Provincia di Roma,

Politico di esperienza e di indiscussa competenza, fu Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la funzione pubblica, sia nel secondo che nel terzo Governo Berlusconi, e seguì in quella veste numerosi provvedimenti, soprattutto per la semplificazione legislativa e amministrativa. fu, insomma, uno dei primi e più convinti sostenitori delle politiche di semplificazione. Per lui il riassetto normativo e la riduzione degli oneri amministrativi costituivano una base necessaria per la competitività del Paese. Il suo impegno in qualità di Sottosegretario è stato apprezzato da tutte le forze politiche, anche di opposizione. Il suo tratto umano si caratterizzava nell'attività istituzionale, come nel privato, per lealtà e disponibilità al dialogo. aveva a cuore la concretezza e poneva al centro del suo impegno politico la risoluzione dei problemi. Quando nella XV legislatura il suo partito passò in minoranza, la sua non fu mai un'opposizione preconcetta e di scontro, ma fu sempre attenta al merito, così come si impegnò sui temi della riforma costituzionale e della pubblica amministrazione. Concluse la sua carriera nelle istituzioni con la nomina, nell'aprile del 2009, a componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e continuò la sua carriera accademica. Saporito, infatti, prima ancora che un politico, è stato e continuò a essere un professore universitario. Eppure, come accademico, ebbe sempre uno spiccato interesse per lo studio dell'organizzazione dello Stato. Pioniere del diritto regionale, ricordiamo le sue monografie sul tema fin dagli anni Settanta. L'ultima monografia, la cui seconda edizione è stata edita nel 2012, ha un titolo evocativo: «Regionalismo, federalismo e interesse nazionale». In questo scritto Saporito, che aveva vissuto il processo di riforma dello Stato in senso federale, affronta con grande lucidità l'evoluzione dei rapporti tra il potere centrale e le e le istituzioni locali, evidenziando il problema e il parametro dell'interesse nazionale. Questo testo è forse una sintesi della sua vita, in cui studio e passione politica hanno sempre camminato insieme. Fu un politico attento all'ascolto, in particolare del mondo della pubblica amministrazione, che in lui ha avuto sempre un costante punto di riferimento. L'umiltà nell'approccio era pari alla competenza e alla capacità di risposta. un politico nel senso più nobile del termine, che diede un prezioso contributo in una fase delicata e di passaggio da un'epoca all'altra del sistema democratico. Il Senato gli rende omaggio ed esprime il suo cordoglio alla famiglia. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo si senta più solo. Learco Saporito veniva dall'Italia meridionale, da Scafati.

capitò di conoscerlo quando, insieme a mia moglie, volli andare qualche giorno a seguire il festival di Spoleto. Aver incontrato una persona amabile, simpatica e festosa come Learco Saporito rese, in quel periodo, meno aspro il mio trasferimento da Napoli a Roma. Siamo stati poi colleghi in questa Assemblea nell'XI legislatura. Saporito era reduce - come lei ha ricordato - da importanti esperienze di Governo con De Mita e Andreotti. Egli era noto ai colleghi parlamentari del Gruppo della Democrazia Cristiana come il massimo esperto, cultore e aggregatore dei dei problemi, delle categorie e delle sottocategorie del pubblico impiego. Eravamo insieme nella 1a Commissione affari costituzionali. Gli emendamenti di Saporito erano un classico dell'attività della Commissione. Il collega Maurizio Sacconi, allora brillante esponente del Governo Amato alla funzione pubblica, e quindi in cerca di razionalità competitiva per l'economia italiana in quei drammatici giorni, si vedeva incalzato da Saporito nella intensissima e generosa ricerca, magari più che della competitività del sistema Italia, della giustizia nel caso particolare. Saporito aveva l'arte di complicare le questioni semplici ma questo - forse io allora non lo capivo era parlamentarismo nel senso più nobile del termine, non meno di quanto Andreotti e l'andreottismo fossero stati semplificazioni di questioni complicate. Insieme a Saporito mi sono trovato, in quella legislatura, a far parte della Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere fu il maestro di vita più importante. Oggi si parla con tante ridicole *technicality* di garantismo e di giustizialismo come se fossero categorie della politologia. Saporito era un punto di riferimento per la sua straordinaria umanità. Non c'era collega raggiunto da un avviso di garanzia e dalla richiesta di autorizzazione a procedere

Learco Saporito, che aveva radici più di sinistra democristiana che di andreottismo o di centrismo degasperiano, con molta coerenza e passione, decise di stare

per portare la storia di Alleanza Nazionale dalla destra verso il centro. Ritornò in Parlamento e al Governo e fu collaboratore, come Sottosegretario, di Frattini prima di Mastella poi e tutti lo ricordiamo, in quest'Aula, come una delle persone migliori e più simpatiche. Mi capitò poi di incrociarlo con la moglie qualche volta nel Sud e qualche volta nell'estremo Nord, a Cortina. Di qui una grande tristezza e un grande affetto del nostro Gruppo per sua moglie e i suoi cari. *(Applausi Signor Presidente, il Gruppo AL-A si associa al dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa del senatore Learco Saporito. Saporito. Il Presidente ha voluto oggi ricordarne la carriera professionale come illustre professore universitario, che ha espletato il suo mandato in tante università d'Italia, come politico legato a questa istituzione, al Senato,

nell'attività politica ma continuava nella vita sociale, con la presidenza dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati. Continuava nella sua attività anche al servizio delle comunità locali, come assessore alla Provincia di Roma,

all'università italiana e alla famiglia che tanto amava. Accanto a questo, desidero ricordare Learco Saporito in modo particolare nel suo ultimo periodo di permanenza parlamentare, quando ho avuto il piacere

interparlamentare, fu tra coloro che ebbero l'idea di creare questo organismo di politica internazionale che rappresentasse i Parlamenti del nostro Mediterraneo, un mare così attanagliato, in modo particolare negli ultimi giorni, da tante situazioni

due esempi importanti di uomini che, nella loro formazione cattolica, trovavano la forza del concetto della politica come servizio per le istituzioni, nelle quali fortemente credevano, e per il proprio Paese, che è un qualcosa che, oggi manca a molti nella politica italiana. Penso che ricordare oggi insieme due grandi galantuomini, due grandi politici e due illustri professionisti dell'università sia un fatto importante importante per questa assise, che è stata onorata della loro presenza. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, ricordo davvero con affetto e rispetto Learco Saporito,

ciò che ha detto poco fa lei, presidente Gasparri, e cioè lo straordinario legame che seppe stabilire con una terra non sua, nel nome del rigoroso servizio parlamentare.

ma che in realtà corrisponde a un'esigenza che dovremmo avvertire maggiormente nella nostra azione politica. il senso dello Stato si traduceva nella dimensione unitaria dello Stato, perché ad esso voleva fosse sempre corrispondente l'unità della Nazione, quell'unità che veniva messa in discussione dai processi disordinati del nostro federalismo, non a caso definito come un albero storto. Ma c'era anche in lui la forte convinzione che lo che lo Stato avesse innanzitutto un dovere di neutralità. Non nascondo - come ha ricordato poco fa il collega Compagna - le nostre forti ragioni di dissenso, un dissenso alto e civile. e civile. Più volte, nella mia esperienza politica, parlamentare e di Governo, ho operato affinché vi fossero un'evoluzione delle amministrazioni pubbliche verso il diritto comune comune e la loro trasformazione dalla prioritaria attenzione agli atti a una maggiore attenzione ai fatti e ai risultati; come nella riforma americana è stato detto, *from red tape to results*. Learco invece sottolineava molto, avendo solide ragioni a questo proposito, la necessità di un agire dello Stato per procedimenti, proprio nel nome della neutralità dell'azione amministrativa, che doveva essere ancor più garantita rispetto alla sua efficacia. Ovviamente tutti e due convenivamo sull'esigenza dell'uno e dell'altro parametro di riferimento, ma inevitabilmente sorgeva il problema di quale assumere per primo. Bene, questo nodo non è risolto. Non è risolto, cioè, il nodo se le amministrazioni pubbliche debbano evolvere - come dicevo - verso il diritto comune e un maggiore orientamento ai risultati e all'efficacia dell'azione amministrativa o se invece le amministrazioni pubbliche debbano ancor più compiutamente rientrare in un alveo pubblico, nell'alveo del diritto amministrativo, nell'alveo di funzioni rigorosamente neutrali rispetto ai cittadini, che mai devono essere sudditi. In questa discussione, che continuerà e forse non avrà mai fine, Learco non sarà con noi, non parteciperà direttamente al dibattito politico e scientifico che continuerà su queste scelte. però, il suo lavoro parlamentare e accademico e attraverso ciò che ci ha lasciato, lui sarà con noi e sarà ancora utile a quella ricerca del bene comune cui ha dedicato tutta la sua vita.

Io non posso che aggiungere - e lo faccio sommessamente, nel senso che non posso venir meno a quello che sento fortemente un dovere

quel naturale segno di essere nato in Campania portava dentro l'azione politica una finta confusionarietà. Quando interloquiva, cercava di sviare l'interlocutore cambiando spesso argomento, ma non perdendo mai di vista l'obiettivo centrale. con me, appena eletto in quest'Aula (venivo dalla Camera e, a quel tempo, si veniva promossi passando dalla Camera al Senato). Incontrai la figura del senatore Saporito, che era Sottosegretario alla pubblica amministrazione, e feci contro il Governo, facendo parte della maggioranza, una guerra per cercare di stabilizzare i precari degli orti botanici di Palermo e Firenze. Presentammo un emendamento; fui, in questo caso, autorizzato dal presidente Schifani, che avevo come presidente del Gruppo e autorevole esponente in Assemblea, a farne un motivo di contrapposizione al Governo e finimmo per sospendere la seduta e andare nella stanza del Governo per discutere di cosa fare di quell'emendamento, che poneva una qualche difficoltà all'Esecutivo, ma che aveva un grande significato locale, sia a Palermo, sia in Toscana (motivo per il quale avevo coinvolto il senatore Mugnai e altri esponenti politici toscani). inframmezzando frasi un po' romanesche, un po' campane, sviandomi dall'obiettivo e cercando di confondermi, mi disse che non era il momento di porre un problema che metteva in difficoltà la maggioranza, fermo nel mio obiettivo di ottenere una cosa che ritenevo giusta. Ne feci non soltanto una questione di principio, ma anche un motivo per potermi, insieme ad altri, astenere sul provvedimento. Rimandammo la cosa di comune accordo e, nel fare ciò, ottenemmo la promessa da parte del Governo che quella disposizione sarebbe stata in seguito approvata. prendendomi da parte, mi disse: «Ma tu, che sei ingegnere, cosa c'entri con l'agricoltura e gli orti botanici?». E ho voluto raccontare il fatto con una certa vanità, perché il personaggio era questo:

mutasse; era già stato Sottosegretario in Governi della Prima Repubblica e, con la sua esperienza, cercava di dare un forte contributo alla politica e al Governo - puntualmente si era informato su quel giovane senatore che poneva una qualche difficoltà. Accanto a quella esternata confusione, metteva una grande precisione nel cercare di superare la difficoltà e di raggiungere l'obiettivo di far votare il provvedimento. un grande personaggio, una persona amabile, puntuale. La reciproca conoscenza e, da parte mia, la grande stima suggellarono nel prosieguo un rapporto del quale mi onoro di essere stato parte e per il quale mi onoro di aver ricevuto l'amicizia del senatore Saporito.

ringrazio per la commemorazione che ha voluto svolgere a livello istituzionale. uomo delle istituzioni, un politico che ha dedicato la propria vita al servizio del Paese, con impegno e dedizione. È stato - come ho testé detto - senatore per ben sei volte, quattro volte con la Democrazia Cristiana e, nel 2001 e nel 2006, con Alleanza Nazionale. È stato uomo di Governo, Sottosegretario alla ricerca scientifica e all'università,

quando fu nominato, dall'allora presidente Silvano Moffa, assessore ai servizi sociali. E l'assessorato ai servizi sociali nella Provincia di Roma era, allora, uno degli incarichi più vicini ai bisogni delle persone. Io ero a quel tempo un giovane consigliere di minoranza che si affacciava alla politica fuori dal proprio territorio, ma ricordo ancora il confronto, il dialogo costruttivo che riuscii a instaurare con Learco, pur partendo da posizioni differenti, benché il terreno su cui affondavano le nostre radici fosse lo stesso. Ricordo le tante volte che ci confrontavamo in Commissione o in Assemblea o le mie visite in assessorato. Oltre a essere sempre ironico e spiritoso,

Di lui ho apprezzato i modi decisi ma cordiali, il suo perseguire il bene comune, il suo vivere la politica non come un fatto personale, ma come organizzazione del consenso per risolvere e migliorare la qualità della vita della gente. questo di lui che voglio ricordare oggi a nome del Gruppo del Partito Democratico. Il suo interpretare la politica e i ruoli a essa connessi come strumento e non come fine, anche da posizioni differenti: questo è l'aspetto che dovrebbe accomunarci. Questo è ciò che resta della nostra esperienza, anche in quest'Aula, come in altre istituzioni, una volta che non ci saremo più. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire molto brevemente in qualità di Presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero,

sempre al di sopra e al di fuori degli schieramenti politici. E, in effetti, era ancora Presidente onorario dell'ANFE. Come senatori del collegio Estero, ma credo come tutto il mondo organizzato e associativo degli italiani all'estero, vogliamo ricordarlo e associarci

Nel 1994 si aprì un dibattito all'interno della destra italiana, dell'allora Movimento Sociale Italiano,

insieme a Fiori, Rebecchini, Armani, Fisichella, Ramponi e tanti altri, che venivano da esperienze politiche diverse - come è stato già ricordato - decise di aderire ad Alleanza Nazionale. importante, la destra, da partito di testimonianza, divenne definitivamente partito di Governo.

(i Costituenti vollero la pena di morte per i casi previsti dalle leggi militari di guerra). Il Parlamento decise di abolirla e, conoscendo la mia totale avversione alla pena di morte di qualsiasi tipo, che avevo sempre sostenuto all'interno

Naturalmente rimase male per quello che gli stavo dicendo, ma reagì con grande dignità e civiltà e non abbandonò mai il partito anche dopo il 2008, seppur non ricandidato. Desidero far pervenire a nome del Gruppo di Forza Italia, alla moglie, ai figli e ai familiari le nostre sentite condoglianze. Non è solo una perdita della famiglia, ma per tutti noi.

Signora Presidente, signori senatori, è la seconda volta che intervengo sul disegno di legge europea, l'ultima è stata nel luglio

ad esempio nella combinazione tra l'articolo 9, sui pacchetti vacanze per i turisti in crociera, e l'articolo 10 sui viaggi degli emigranti. Non mancavano - ripeto oggettivamente comici: ad esempio, la fondamentale normativa che disponeva in ordine al fatto che i camini non potessero essere fatti in materiale infiammabile, e via legge è oggettivamente meno tragico, il che è positivo, ma è drammaticamente comico. Faccio un elenco dei fondamentali contenuti presenti nel testo del Governo (è evidente che gli emendamenti dal Parlamento sono a margine): stiamo votando un testo che contiene norme sull'etichettatura dell'olio e del miele; norme relative all'IVA per il basilico, rosmarino e salvia fresca; norme relative all'IVA per i preparati per il risotto; norme relative alla raccolta dei tartufi norme relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma (cosa voglia dire francamente non lo so, ma suppongo che sia stata fatta oggetto di approfondita riflessione da parte del Governo) e molto altro. Credo che in questo testo ci sia, a valle, il riflesso della struttura della legislazione europea.

151 metri lineari, più o meno 150 divine commedie. Questo tipo di produzione legislativa ha caratteri oggettivamente demenziali, perché mai nella storia si è configurato un organismo legislativo così produttivo credo anche fortemente illegale. La struttura costituzionale europea prevede il riparto delle competenze, conservate dagli Stati, devolute al superiore livello dell'Unione e concorrenti. Sulle competenze concorrenti dovrebbe giocare il criterio previsto nel Trattato della sussidiarietà, definita attraverso uno specifico protocollo. La sussidiarietà vuol dire che fai sopra solo quello che non puoi fare ugualmente bene sotto. Ma voi pensate che sia nella logica costituzionale costituzionale europea la disciplina fatta sopra, ma recepita sotto, sul miele? Trovo che ciò non solo sia la prova di elementi demenziali della struttura europea, ma anche di elementi illegali. Siamo in totale violazione della norma del trattato che prevede la sussidiarietà: si fa a livello di Stato tutto ciò che si può fare a livello di Stato, e sopra, solo per eccezione, solo quello che meglio si può fare a livello di Unione. L'eccezione, in una logica leviatanica e assolutistica, è diventata la regola, tanto che qui stiamo applicando norme che discendono dall'alto estese su un catalogo infinito di contenuti: l'esatto opposto dell'eccezione. A me è capitato di sentire in questa sede il Presidente del Consiglio, da una parte, ironizzare contro i burocrati europei, dall'altra parte (ed è oggettivamente

alla normativa europea. Siccome il cumulo delle cariche non è vietato, mi chiedo se siano più stupidi i burocratici o più stupidi quelli che da una parte attaccano i burocrati e dall'altra si vantano di aver assecondato, con Grazie. l'ironia, è in realtà drammatica. Siamo alla fine della struttura europea: se l'Europa è questo, posso capire che le *élite* - *élite* si fa per dire - più o meno cosmopolite o strampalate

Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Silea, in provincia di Treviso. Benvenute e

discussione. Il disegno di legge oggi alla nostra attenzione, che il Governo ha presentato lo scorso 3 febbraio, si inserisce in un percorso responsabile e laborioso, portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti. Il dato positivo è che le procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono in diminuzione. Difatti, il numero delle procedure scende a 80, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Inoltre, sempre la Commissione europea, ha disposto l'archiviazione di due casi EU Pilot già chiusi negativamente, che avrebbero potuto presto dare origine a procedure di infrazione. Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quindi eterogenei, sia per materia che per competenza. Questo, tuttavia, deve farci comprendere bene come le decisioni europee - in tutte le loro discutibili forme - incidano nella vita politica, sociale ed economica del Paese e nelle nostre vite quotidiane: ne sono un esempio le direttive i cui contenuti incidono sulla salute, sull'alimentazione, sulla libera circolazione, come anche in tema di giustizia. Non a caso, la conformità del diritto comunitario con il diritto interno - ferma restando la gerarchia delle fonti - ha la duplice funzione da una parte di adeguare la legislazione dei singoli Paesi membri e, dall'altra, di elevare sempre di più gli *standard* qualitativi dei cittadini europei. Credo che questa funzione positiva dell'Unione europea molto spesso venga dimenticata e, invece, andrebbe più correttamente valorizzata. Come accennavo, comunque, considerata la diversificazione delle materie contenute, concentrerò il mio approfondimento sul Capo VII, contenente disposizioni in materia di energia, non solo perché me ne sono occupato in Commissione politiche europee, ma soprattutto perché anche a livello internazionale si è arrivati finalmente a una consapevolezza sul tema. Vale la pena ricordare che lo sviluppo della politica energetica europea è dovuto essenzialmente a due ragioni: da un lato deriva dalla frammentarietà della competenza energetica, con l'assenza di una base giuridica unica e generale nel Trattato dell'Unione europea

Il percorso del diritto europeo dell'energia si è delineato attraverso un sistema di espansione delle competenze materiali dell'Unione, che, più in generale, è un tratto rilevante del dinamismo evolutivo del diritto dell'Unione. Nondimeno, la competenza energetica dell'Unione si sviluppa attorno ad un nucleo storico della normativa *antitrust* in campo energetico, laddove sono emersi ulteriori profili della disciplina energetica, che incidono sulla tutela ambientale e sulla tutela della sicurezza energetica. La combinazione di obiettivi di tutela della concorrenza, protezione dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ha creato il problema dell'individuazione della corretta base giuridica, ovvero dell'ammissibilità di atti energetici adottati adottati su un doppio fondamento normativo, ovvero quello nazionale e quello comunitario. Per questo l'esercizio della competenza sull'energia è da sempre un elemento fondamentale della politica economica e industriale di uno Stato. Nel campo delle relazioni europee e internazionali, essa assume un connotato ancora più decisivo poiché diviene un elemento di stabilizzazione nonché uno strumento strategico per assicurare la competitività dei sistemi economici. Analizzare, quindi, la dimensione giuridica della politica energetica europea vuol dire filtrare, dall'insieme eterogeneo di elementi che riguardano la regolamentazione dell'energia, anche aspetti che hanno un impatto, diretto o indiretto, sul diritto dell'Unione. Non sottovalutabile, poi, il fatto che la legislazione europea affida ai regolatori nazionali importanti responsabilità in tema di tutela dei consumatori, promozione di prezzi equi e introduzione di strumenti semplici per esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore e per la risoluzione delle controversie. Ne conviene, perciò, che i problemi giuridici relativi alla disciplina del settore energetico sono essenzialmente connessi alla separazione di competenze, diritti e responsabilità tra l'Unione e gli Stati membri: la ripartizione della competenza energetica si muove all'interno di un processo in evoluzione, ancora lontano da una sistematizzazione definitiva. Nello specifico, l'articolo 28 reca disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Difatti, già la legge n. 96 del 2010, ovvero la legge comunitaria 2009 (Atto Camera 2449), aveva delegato il Governo al recepimento della direttiva n. 72 del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica e della direttiva n. 73 del 2009 dal decreto legislativo n. 93 del 2011, si ponevano gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti vulnerabili. Ciò premesso, le valutazioni nel merito dimostrano che un mercato europeo pienamente funzionante dovrebbe consentire all'energia elettrica di circolare liberamente dove è più necessaria, richiesta e valutata, di trarre il massimo vantaggio dalla concorrenza transfrontaliera e di fornire i giusti segnali e incentivi per orientare correttamente gli investimenti. Inoltre, si dovrebbe garantire che l'energia elettrica sia distribuita unicamente in base ai segnali del mercato. Tuttavia, allo stato attuale, non è sempre così. Mentre l'accoppiamento dei mercati, dove è stato applicato, ha comportato una maggiore correlazione tra i prezzi all'ingrosso, il valore assoluto dei prezzi differisce in modo significativo anche nei mercati vicini e i differenziali dei prezzi non si contraggono. Gli adeguamenti normativi contenuti all'articolo 28 in fase di *iter* parlamentare in Commissione - condivisibili e necessari - dimostrano tutta l'attenzione del legislatore per colmare lacune e diverse interpretazioni attuative delle direttive n. 72 e 73 del 2009: in particolare sono state chiarite le relazioni tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, nonché il fine ultimo di salvaguardare il valore dell'indipendenza e della discrezionalità degli organi regolatori rispetto alla pubblica amministrazione alle dipendenze dell'Esecutivo nazionale. Inoltre, altrettanto condivisibili sono i correttivi interpretativi contenuti nel comma 2 che modificano l'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, laddove vengono ribaditi gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori ponendo maggior efficacia sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione era stata demandata ai singoli Stati membri. Il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi periodi critici, fa sì che saranno garantiti non solo i diritti e gli obblighi relativi alle forniture ma anche misure di tutela ai clienti finali nelle zone isolate. Meritevole è, quindi, alla luce della richiesta europea, la sostituzione dell'attributo «vulnerabili» con quindi ora si parla di utenti protetti. In conclusione, la riflessione che spero sia condivisibile da tutta l'Assemblea, è che i cittadini europei non sono oggetto solo di vincoli - che io per primo riconosco talvolta restrittivi e stringenti - ma anche destinatari di crescita e sviluppo per una qualità della vita migliore.

Signor Presidente, signore e signori senatori, rappresentanti del Governo, come è a conoscenza anche di quest'Assemblea, diversi sono gli oneri derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea. Tra questi, quelli regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, tra cui per l'appunto la cosiddetta approvazione della legge europea, attraverso la quale cui si dovrebbe periodicamente adeguare l'ordinamento interno, ponendo rimedio alle sanzioni che troppo spesso sono state comminate all'Italia per i ritardi o le omissioni nell'adeguamento alle direttive e ai regolamenti europei. Inoltre è risaputo che dal 2008, con il meccanismo EU Pilot, si è costruita

- mi si consenta - di una classe politica che ha creduto che in Europa si potesse continuare a fare interessi di bassa bottega, non diversamente da come si faceva nei propri confini. Una classe politica che spesso - quando ci andava - ha considerato Bruxelles una gita di piacere, piuttosto che il luogo decisivo dove rappresentare e tutelare in ambito comunitario diritti, doveri e interessi del popolo italiano. I 22 articoli di cui è composto il disegno di legge in esame intendono chiudere due procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot, nonché sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato. I settori interessati sono vari e, pur non volendo attribuire in modo pretestuoso all'attuale Governo tutte le responsabilità in ordine ai casi in cui il disegno di legge in esame dispone interventi (anche perché le maggiori responsabilità sono da attribuire a chi abbiamo mandato in Europa), di fronte a un Esecutivo rinunciatario, soprattutto in alcuni dei casi EU Pilot in cui si prosegue sulla strada dell'ossequio alle indicazioni della Commissione, senza tenere il punto a difesa degli interessi dei cittadini italiani. Ci sono ambiti in cui abbiamo tutte le ragioni per contrastarne le decisioni, in quanto ancorati a principi europei ancora maggiori di quello del libero scambio e che sono a fondamento dell'esistenza stessa dell'Unione europea, quali la trasparenza e la corretta informazione ai cittadini.

che non sanano sanzioni, ma intervengono su casi EU Pilot che vanno a limitare i valori che ho indicato. I primi tre articoli, su cui ho presentato emendamenti soppressivi che invito a votare, denotano infatti un atteggiamento rinunciatario che questo Governo continua a tenere proprio nel settore agroalimentare, che dovrebbe invece costituire il vanto internazionale del nostro *made in Italy*, pure celebrato in pompa magna con il recente Expo. L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, risolve il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo,

e libera concorrenza. Alla lettera *b)*, poi, si è intervenuti per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura, questa volta del miele,

Sul miele, la norma italiana che questa legge va a modificare prevede, per le confezioni importate da altri Stati membri di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Infine, l'ultimo articolo su cui mi sono soffermato, l'articolo 3, riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari. È il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. consumatori. La nostra norma, su cui ora si vuole intervenire, definisce come Paese d'origine del prodotto il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Questo contrasta - così ci viene a dire la Commissione europea - con il regolamento n. 1169/2011, che stabilisce invece che il Paese d'origine del prodotto sia quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale. Mi chiedo perché cedere senza combattere a degli EU Pilot interessati della Commissione europea, quando risulta di lampante evidenza come ognuna delle norme citate sia ispirata alla tutela delle ragioni del consumatore, anzi di un consumatore evoluto (quale è quello italiano), e sia rispettosa di un altro principio fondamentale in una democrazia, non solo alimentare, che è quello delle esatte informazioni, anche a tutela della salute. Si tratta di norme ispirate alla trasparenza, quale strumento indispensabile del consumatore ed in genere del cittadino per effettuare una scelta consapevole, norme che provengono dall'esperienza, perché spesso alla mancata segnalazione del Paese d'origine della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione dei prodotti si accompagna l'ingannevole presenza di marchi o segni distintivi italiani caso del Parmesan), che inducono ad individuare nel nostro Paese la reale origine del prodotto; sono quindi norme che contrastano la contraffazione. Si tratta di norme ispirate dal buon senso di un popolo, il nostro, che è all'avanguardia nella produzione e nel consumo di qualità; norme il cui carattere preventivo è in grado di rappresentare l'unico e solo freno alla sofisticazione alimentare di massa ed al *trash food*, della quale è evidente che certa industria interessata si vuole fare paladina. È evidente, ed emerge da da ogni autonoma indagine delle associazioni dei consumatori, come le norme minime che provengono dall'Europa sulla qualità delle produzioni agroalimentari stiano abbassando sempre di più la tutela dei consumatori europei, anche dal punto di vista della salute. E noi, che facciamo vanto dei nostri prodotti IGP e DOP, saremo - temo - fortemente penalizzati se non difenderemo con le unghie e con i denti le nostre produzioni di qualità. Chissà poi cosa accadrà nelle more dell'approvazione del famoso TTIP. La qualità della vita e la salute non possono essere sacrificate sull'altare dei principi economici e dei profitti che si nascondono dietro la cosiddetta liberalizzazione del mercato e delle merci, se non mediati - così come

che le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione sarebbero complicate per il nostro Paese e ci costringerebbero a difenderci davanti alla Corte europea. Ma, se non lo facciamo ora e su questi temi, quando lo faremo? Si tratta sono sicuro - sui quali il Governo avrebbe tutto il sostegno del Parlamento e del Paese e che il presidente Renzi potrebbe sfoggiare con orgoglio - questa volta sì, a ragione - in tutte le sedi europee e a nome di tutto il popolo italiano.

Presidente, ho fatto parte della 14a Commissione per più anni - poi sono passato ad altra Commissione - e so benissimo quanto sia importante e determinata, e come sia ben guidata, con moderazione e serietà, dal presidente Vannino Chiti. cosa emerge anche questa volta? Già la prima volta (fui io relatore sulla legge di delegazione europea) approvammo la norma che riguardava

Abbiamo già pagato 150 milioni di euro per la mancata bonifica delle discariche, per quelli che sono stati considerati aiuti di Stato a Chioggia e Venezia e per alcune norme sulla formazione-lavoro, e tante altre condanne incombono su questo Paese. C'è un'Unione europea che comunque,

Ci apprestiamo anche a subire salassi incredibili per il problema degli impianti depurativi delle acque reflue. È un salasso su cui la Corte di giustizia sta per pronunciarsi, che sarà enorme se non ci difendiamo nel modo dovuto. È tutto un paradosso, perché abbiamo circa 3,2 miliardi di euro stanziati per queste opere, ma non è stata fatta da anni nemmeno una gara e tutto e tutto passa nel silenzio degli enti locali e delle Regioni. È una cosa incredibile, assurda. È vero che bisogna adeguare le tariffe rispetto alle acque reflue, ai depuratori e a tutto il resto,

Perché non devono essere chiari i quantitativi di olio acquistati e quelli immessi sul mercato? Perché dobbiamo permettere che venga immesso sul mercato olio adulterato? Questa è la realtà.

Perché dobbiamo demandare ai produttori l'indicazione dei termini di scadenza dell'olio (ha dell'incredibile), demandando loro la responsabilità e giocando sulla pelle dei consumatori? Sono cose che non si riescono assolutamente a capire. Su questo c'è la carenza totale di un'azione di governo e di presenza. Sulla etichettatura continuerò sempre a insistere (vale per l'olio e per altri prodotti): perché no? Perché non si deve controllare ciò che viene acquistato e quanto viene prodotto? Siamo complici di chi e di che cosa? Perché continuiamo a distruggere tutti i nostri produttori di latte, che devono vendere a 29 centesimi,

queste norme possono essere anche fatte, ma così - lo evidenziava anche il senatore Molinari - ci vuole un po' un atto di coraggio. Ci rendiamo conto delle difficoltà e delle responsabilità cui andremo incontro?

Questa è la realtà che abbiamo, e diventa quasi assurdo ciò a cui assistiamo: il nostro rincorrere situazioni spesso assurde; il nostro non essere capaci di risolvere problematiche interne, come quelle delle acque reflue e dei depuratori; la nostra incapacità di difendere ostinatamente tutto ciò che è prodotto italiano, non difendendo i nostri produttori e tutto il resto;

siamo capaci di difendere tutto ciò che è la nostra agricoltura. L'agricoltura italiana muore a favore dell'agricoltura francese, tedesca e spagnola: questo è il dato reale, ma noi non facciamo assolutamente nulla. Per questo motivo e per quelle poche cose che si sono potute dire in dieci minuti certamente il nostro voto non sarà il massimo dispiacere. Ma è arrivato il momento di mettere un punto fermo. L'Italia in questa Europa, per quanto mi riguarda, ci sta volentieri, ma se l'Europa è solo matrigna allora non ci si può più stare. So che è una parola grande, ma spesso la colpa è nostra: la nostra incapacità di difendere Non è possibile, sinceramente. Un po' di coraggio, un po' di amor patrio - non deve sembrarvi una parola superata dai tempi - è ciò che manca. L'italianità dove sta? sta? Gli altri invocano dalla mattina alla sera, e noi cosa stiamo invocando? Ciò che è giusto, ciò che è nostro, la nostra qualità. Ma non facciamo nulla per difenderla. È qualcosa di incredibile che sinceramente ci lascia sconcertati. Non sono certamente un ragazzino, ma vedere la discesa di questo Paese rispetto alla propria identità ha dell'incredibile, non veder difendere la nostra ricchezza naturale e vederla sempre più depauperata, chinando la testa rispetto agli altri *partner* europei, come la stiamo chinando anche in altre cose (poi ne parleremo). Vediamo come ci salutano Francia e Germania rispetto ai loro stretti interessi. Noi dovremmo essere quelli sempre aperti al mondo; loro più ricchi di noi e noi sempre aperti a loro: non è possibile. Difendiamo ciò che è giusto, ciò che è nostro,

giustificare i ritardi del passato. Quindi si modificano i titoli delle leggi per dire che tutto è a posto: una tecnica ormai collaudata da parte del Governo Renzi. L'importante è che la copertina, quello che sta scritto sopra al testo di legge, sia convincente. Se poi quello che sta dietro è totalmente vacuo, vuoto, non esiste addirittura, chi se ne importa; l'importante è che parta il *tweet*, che la gente si rassicuri e che tutto il messaggio vada a destinazione. visto che il presidente Renzi si è abituato anche ad aspetti mediatici, iniziamo questa discussione generale sull'Unione europea, ovvero sulla legge europea 2016, con due immagini contrapposte e parallele, specchio dello stesso Governo.

Presidente del Consiglio dei ministri e Alto rappresentante per la politica estera europea, colei per il quale il Paese ha politicamente versato sangue perché Renzi ci ha fatto rinunciare a posizioni chiave per poter avere questa figura in Europa che doveva tutelare gli interessi dell'Italia. Presidente, questo articolo d'inchiesta partiva da una considerazione semplice: quali sono le azioni fatte dalla ministra Mogherini nell'Unione europea? Cito e leggo testualmente: «È stata lei, lo scorso settembre, a proporre di concedere alla Tunisia quote extra di olio di oliva esportabile esentasse nell'Unione europea». Complimenti. Con i voti poi del Partito Democratico, costei ha inserito nel mercato europeo 70.000 tonnellate di olio tunisino. della cooperazione e perché bisogna aiutare la Tunisia perché altrimenti viene aggredita dall'ISIS. Ma cosa c'entra? Stiamo parlando di un Paese che non difende i propri interessi commerciali.

darci una risposta a quello che scrive la Confederazione generale dell'agricoltura il 21 marzo. Essa si rivolge a lui, ai componenti della Commissione agricoltura e agli altri parlamentari europei dicendo di fermarsi, perché con quello che stanno facendo, introducendo queste tonnellate di olio d'oliva

Che senso ha l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea se non è nell'interesse dell'Italia stessa e degli europei? Questa domanda verrebbe da porsi. Certamente dalla lettura di questo provvedimento ne esce un'immagine

cose sulle quali il Governo, anziché iniziare una dura battaglia in sede europea, non batte ciglio e semplicemente si adegua perché ce lo chiede l'Europa. Mi piacerebbe avere il ministro Martina a rispondere di queste cose, ma evidentemente un conto è la realtà narrata, un altro invece sono i fatti, rispetto ai quali il ministro Martina scappa. Presidente, nel provvedimento si parla dell'aumento dell'IVA sui preparati per risotto e per coprire una differente tassazione sul gioco d'azzardo. d'azzardo. Presidente, si parla anche delle obbligazioni alimentari in materia matrimoniale. Si parla della tassazione dei veicoli degli studenti europei in Italia,

in aumento). Come farsi mancare anche una norma specifica in merito ai tartufi? Inoltre il provvedimento reca raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di disposizioni relative alla natura della fauna selvatica omeoterma. Questa è la ragione per la quale partecipiamo all'Unione europea. Quant'è lontana quell'Unione europea di Adenauer, di De Gasperi, di Schuman! Non c'entra niente. Questa è una melassa di burocrazia e di regolamentazione che tutto ingrigisce, alla quale noi vorremmo invece un'azione del Governo forte a tutela dei nostri prodotti, che sono anche *made* in Europa, perché nel momento in cui un prodotto è *made in Italy,* significa qualità anche per la stessa Europa. invece, si gioca al contrario: bisogna annientare il prodotto *made in Italy*, affinché coloro che commerciano e non producono possano smerciare i loro prodotti di bassa qualità

Ne dovremmo parlare per ore, signor Presidente, ma temo che sui giornali troveremo solo trafiletti, perché raccontare questa realtà di Europa

tra cui in particolare quello riguardante la produzione e la commercializzazione dell'olio d'oliva e quello del comparto vitivinicolo. Abbiamo letto in queste ore il contenuto del trattato TTIP, i cui negoziati vengono portati avanti in segreto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

che si impegnerà a dare veloce attuazione a questo tipo di regolamentazione commerciale. No, signor Presidente, noi ci opporremo, perché è in gioco non solo la salute dei cittadini, ma anche la stessa esistenza dei nostri cittadini in quanto produttori, consumatori e in quanto cittadini italiani prima ancora che europei.

onorevoli colleghi, con il generico titolo «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015», l'Europa, nei fatti, assesta un duro colpo sia ai nostri agricoltori, che ai nostri consumatori. Da tempo questa non s'è dimostrata essere l'Europa dei popoli che auspicavano i nostri Padri fondatori, bensì un'Unione europea che strizza l'occhio ad una finanza incontrollata, a politiche massacranti per i milioni di cittadini europei, ma non per le poche multinazionali mondiali alle quali stende tappeti rossi. Il forte aumento delle disuguaglianze avvenuto nel corso degli ultimi trent'anni nei maggiori Paesi capitalistici può infatti essere individuato come la causa ultima della crisi economica in corso. La stagnazione o il declino dei salari reali, in tutti i casi la loro persistente tendenza a non tenere il passo con gli aumenti della produttività del lavoro, hanno fatto sì che gli aumenti del reddito totale che di anno in anno si verificavano nelle principali economie affluissero al ceto più benestante della popolazione, tendendo ulteriormente a concentrarsi al suo interno nei sottogruppi più ricchi. Gli effetti depressivi sui salari sono i più ovvii e si traducono per le economie più sviluppate in un'offerta di lavoro a basso prezzo praticamente illimitata. Anche quando si tratti di manodopera scarsamente qualificata, l'impatto del fenomeno non resta circoscritto ai livelli più bassi della scala delle retribuzioni, ma impatta fortemente su tutta la forza lavoro. La Germania, Paese forte dell'Unione, guida di fatto la politica della BCE. Dappertutto in Europa i Governi persistono nel ricorso a politiche di austerità consistenti in tagli allo Stato sociale e ai servizi pubblici essenziali. Malgrado si riconosca apertamente che tali politiche causeranno nei prossimi anni cadute sensibili dei livelli di attività, si afferma però che esse non mancheranno alla fine di assicurare la ripresa di un processo di crescita stabile. Ce lo chiede l'Europa! Ci sentiamo continuamente dire: «Il sistema bancario è solido e privo di rischi» (così Padoan nell'ottobre 2014). Oggi invece Padoan dice: «Serve più borsa, valutare un fondo monetario europeo con risorse del MES». Come fidarsi di questa Unione europea che è nelle mani una Commissione di esecutori dell'alta finanza che esprime una politica di trattati commerciali come se fossero note a margine di un ufficio di periferia? Come fidarsi di una Unione europea che afferma di aver ricevuto dai 28 Governi un mandato di protezione dal quale non deve derogare? Non fidarsi è imperativo. Ogni volta che abbassiamo le difese si aggiungono errori nei confronti degli Stati e dei nostri interessi, nel nostro caso soprattutto nel settore dell'agricoltura, comparto ormai devastato da accordi e da disposizioni capestro. Uniformare le indicazioni di origine sulle etichette dei produttori di miscele di olio di oliva, del miele e delle materie prime agricole, perché la Commissione europea ritiene discriminatoria e non armonizzante in materia di leggibilità, accresce la differenza tra chi rispetta le regole della qualità del prodotto e chi non ce la fa. Così si rischia di livellare al ribasso, e di non premiare le eccellenze. La ricerca di protezione del consumatore viene relegata cosi al signor mercato e non più allo Stato, demandando la competenza del controllo del prodotto, sapendo bene quanto il mercato globale al quale ci stanno abituando, abbia solo la logica della massima tutela del profitto e scarsamente della tutela della qualità. Si continua quindi, ancora una volta a fornire ossigeno allo spettro della globalizzazione livellante. colleghi, è indiscutibile che l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea comporti per noi degli obblighi cui dobbiamo giocoforza ottemperare. Sappiamo pure che questo testo trova la sua *ratio* nella necessità di impedire che nei confronti dell'Italia vengano aperte procedure d'infrazione. Tuttavia, si impone una riflessione - come già evidenziato dai colleghi intervenuti sulla necessità che l'ottemperare agli obblighi europei non possa e non debba diventare una supina e acritica accettazione di regole che, intervenendo in maniera importante sul nostro tessuto produttivo, rischiano poi di rivelarsi particolarmente dannose. Da più parti in quest'Aula si è visto l'impegno profuso da tanti parlamentari nella difesa del *made in Italy*, nella difesa di un *brand* che, concettualmente, nel mondo è indice di qualità e di serietà produttiva. produttiva. In un momento in cui i consumatori sono sempre più preoccupati per l'invasione di prodotti, specie agricoli ed alimentari, provenienti dai Paesi esteri (di cui non è ben chiara l'origine, né i protocolli di produzione e di coltivazione, né la tracciabilità), in un momento in cui la domanda di tutela alimentare diventa sempre più forte, credo sia doveroso da parte nostra stimolare e sollecitare il Governo a porre in essere con la Commissione europea un'interlocuzione più forte e più incisiva, che non faccia sconti sulla necessità di tutelare i cittadini italiani, non solo sull'autenticità dei prodotti che acquistano, ma anche sulla consapevolezza e sulla veridicità delle informazioni che riguardano i prodotti che arrivano sui nostri mercati. Per quanto riguarda le disposizioni riguardanti la filiera degli oli di oliva vergini, ad esempio, prendiamo atto che il testo che stiamo esaminando prevede certamente che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva deve essere stampata in un punto evidente, tale da essere «visibile, leggibile e indelebile, non nascosta né oscurata o limitata» e tuttavia non possiamo non dire che viene soppressa quella «più evidente rilevanza cromatica», presente nella legislazione interna, che invece aiuterebbe il consumatore a focalizzare immediatamente l'origine dell'olio e magari orientarlo verso l'acquisto di un prodotto italiano, sulle cui qualità e sul cui controllo magari facciamo maggiore affidamento. Il problema è quello dell'adeguamento della vigente disciplina interna alla normativa europea. Sulla questione è intervenuta la Commissione europea, la quale ha sostenuto che l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità. Mi viene da dire che per l'Europa il principio di concorrenza per l'industria finisce per essere prevalente rispetto alla necessità che l'acquisto da parte del consumatore di un bene alimentare così importante come l'olio di oliva sia sempre più consapevole. Come dire, privilegiamo gli interessi dell'industria rispetto a quello dei cittadini e dei consumatori. Ma lo stesso si potrebbe dire per le disposizioni relative all'etichettatura del miele. Anche in questo caso l'Italia è stata oggetto di formale richiamo da parte della Commissione europea per quanto riguarda l'etichettatura del miele. Il caso è stato originato da alcuni sequestri amministrativi di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica dizione «miscela di mieli originari e non originari della CE», al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Ci è stato formalmente contestato di aver reso obbligatoria l'indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione, andando oltre a quanto stabilito dalla normativa europea. Con l'articolo 2 di questo disegno di legge l'Italia è chiamata a sanare il caso richiamato e si chiarisce che, nei confronti di mieli prodotti in altri Stati membri

le esigenze del nostro Paese che non possono cadere in uno stato di soggezione e in un atteggiamento di quasi rassegnazione rispetto alle cose che vengono decise oltralpe. *(Misto-Idv)*. Il capo VIII della legge europea 2015 contiene disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva n. 80 del 2004. La suddetta direttiva si propone di garantire alle vittime di un reato intenzionale violento un risarcimento equo ed adeguato per i danni subiti, a prescindere dal luogo - all'interno dell'Unione europea, ma

di qualsivoglia misura di attuazione e conclusasi con una sentenza di condanna. Le misure previste dal provvedimento sono state ritenute però non del tutto adeguate dalla Commissione europea. Il decreto legislativo del 2007, infatti, non ha proceduto alla istituzione di un comprensivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reato, ritenendo adeguati i sistemi di indennizzo e risarcimento contemplati già dall'ordinamento per alcune tipologie di reato (quali quelli di stampo mafioso o terroristico) e non, invece, estendendo il sistema nazionale d'indennizzo a qualunque fattispecie di reato qualificabile. Ancora, la questione relativa alla parziale trasposizione della direttiva 2004/80/CE è emersa anche a livello nazionale, ove si sono registrati due divergenti orientamenti giurisprudenziali quanto alla possibilità di ottenere un simile risarcimento in casi concernenti cittadini residenti in Italia e vittime di reati commessi sul territorio italiano, ovvero in assenza di un elemento di transnazionalità. In sostanza, l'Italia ha recepito questa direttiva solo in parte, cioè solo per la parte relativa ai reati transfrontalieri, ovvero qualora il reato sia consumato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima.

che, una volta uscita dall'ospedale, dovrà andare a stare in una sorta di struttura - simile ad un ospizio, diciamo così - insieme ai malati di Alzheimer, che nulla hanno a che fare con la patologia di Chiara. Chiara è totalmente a carico del padre, il quale ovviamente non potrà garantire alla figlia, ridotta come un vegetale, il sostegno enorme di cui necessita, godendo della sola indennità di accompagnamento oggi riconosciuta a Chiara;

Nello specifico, l'indennizzo a carico dello Stato, riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, deve essere equo e adeguato, al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima e non solamente elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. L'indennizzo dovrebbe essere corrisposto anche qualora la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura

qualora sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti. Il testo in esame, invece, sul punto prevede che l'indennizzo venga corrisposto qualora la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto. A ben vedere, però, in tal modo vengono limitate le ipotesi di risarcimento, così come rappresenta un restringimento, che si auspica venga eliminato, la condizione per la quale la vittima debba essere titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a

danno. Nel capo VIII in esame viene previsto che la domanda di indennizzo sia presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita. Al riguardo, ritengo invece che la domanda debba essere presentata generalmente entro il termine prescrizionale di cinque anni. Infine, il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime non dovrebbe costituire, così come previsto all'articolo 32 della legge europea in commento, una parte del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,

fase emendativa. Questa legge può darci la possibilità di rispondere in maniera più concreta ai danni patiti da molte donne vittime di violenza. Ovviamente l'indennizzo che potranno ricevere non cancella e non annulla il danno subito ma può aiutare ad affrontare un percorso di ricostruzione personale e reinserimento in una vita normale. capitolo a parte merita, poi, il discorso relativo alla necessità di mettere in atto una serie di atteggiamenti al fine di prevenire il femminicidio, che continua purtroppo ad avere numeri molto alti nel nostro Paese, nonostante sia un Paese democratico ed erudito

terziario che si è determinato frequentemente per estrapolazione da più complesse società produttive di beni o di servizi e che, in ragione di tale faticosa estrapolazione, ha dato luogo anche a meccanismi di forte inefficienza. La proposta del Governo, che trae spunto da una sentenza della Corte di giustizia europea, vorrebbe classificare tutti i cambi di appalto come cessioni di ramo d'azienda, con la conseguenza della piena continuità di tutti i fattori d'impresa e di tutte le posizioni,

quanto siano necessarie non solo le attività tese a superare le gestioni dirette da parte delle pubbliche amministrazioni locali ma appalti che appalti che privilegino proposte di discontinuità rispetto alla presente inefficienza, proposte cioè caratterizzate da alti livelli di efficienza, così da ricondurre lo stesso trasporto pubblico locale nell'ambito nell'ambito di attività performanti che non consegnano, come oggi accade, continua accumulazione di debito pubblico. La sentenza da cui muove la proposta del Governo atteneva peraltro proprio al trasporto pubblico locale e il suo dispositivo conclusivo ci ha detto che, ove gli elementi materiali contribuiscano in maniera importante all'esercizio dell'attività, l'assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore di un livello significativo di tali elementi che sono indispensabili

non è applicabile in assenza di cessione di elementi materiali significativi tra il vecchio e il nuovo appaltatore. Non si comprende allora come la proposta del Governo consista in una modifica radicale della legge Biagi, che ricordo disponeva che in ogni caso i cambi di appalto non rappresentano cessione di ramo d'azienda. Quella affermazione era probabilmente eccessivamente rigida e tuttavia ora verrebbe sostituita, con l'abrogazione della norma stessa, con un implicito riconoscimento che ogni cambio d'appalto finisce, al contrario, per costituire cessione di ramo d'azienda. Ho descritto prima la conseguenza principale che ne deriverebbe in termini di prosecuzione indefinita di condizioni di complessiva inefficienza nella gestione di attività di servizio. Aggiungo anche quella specifica di un appaltatore marginale che perde l'appalto e che, con esso, potrebbe cessare la propria attività. sarebbe legittimato a scaricare sul nuovo appaltatore il mancato pagamento di tutti i salari e contributi ai lavoratori in forza della responsabilità solidale che conseguirebbe alla qualificazione del cambio di appalto come cessione di ramo d'azienda. La mia proposta è pertanto quella di una regolazione più coerente con la sentenza europea da cui

si consideri l'eventuale presenza di elementi di discontinuità che determinino una nuova identità di impresa. In questi casi l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non può costituire trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, proprio come conclude la

materiali di impresa, è condivisa dalle parti sociali. Mai nel dibattito interno alle istituzioni o alle parti sociali si era sollevato il problema oggi

il genuino cambio di appalto e - invece - il mero trasferimento d'azienda o di parte di essa, indicando gli elementi di discontinuità,

Va ricordato che il disegno di legge in esame si prefigura come un atto di recepimento un po' canaglia e sicuramente creativo, come solo questa classe politica sa fare,

agli articoli 1 e 3), perché c'è una fase molto lunga prima di entrare effettivamente in infrazione. Dopo vorrei concentrarmi sul perché il Governo abbia deciso di recepirli proprio ora. Ricordiamo inoltre che l'Italia è in procedura di infrazione ed ha quattro condanne, due che riguardano gli aiuti di Stato e due che riguardano invece la gestione innominabile dei rifiuti in generale e in particolare in Campania, sulle quali mi pare che questo Governo non stia facendo assolutamente nulla, per cui queste procedure di infrazione sono di fatto accettate e le stiamo pagando. allora: perché andare in procedura di infrazione su questioni che danneggiano la salute dei cittadini e invece non cercare di contrattare ancora per un po' su questioni che danneggiano il *made in Italy*? del contenuto di questa legge, vorrei aggiungere un altro elemento di metodo, sicuramente discutibile, con cui è stata elaborata questa legge europea. Molti degli articoli presenti nella legge sono stati aggiunti successivamente e non sono passati dalle Commissioni competenti. Quindi, oltre alla secretazione degli oggetti per cui siamo in infrazione e oltre alla scarsa discussione in Commissione, ci sono articoli che le Commissioni competenti non hanno potuto esaminare e che quindi sono stati introdotti in maniera surrettizia e successiva solamente in 14a Commissione. Credo che questo sia un fatto molto grave, perché i provvedimenti devono essere prima valutati nel merito dalla Commissione competente. Un altro elemento di metodo è il fatto che molti dei nostri emendamenti sono stati bocciati, in base all'articolo 81, non perché provocavano ma perché - come ha detto la Commissione bilancio - ci sarebbe stato il rischio di andare in infrazione. Anche questa è una vergogna, perché è chiaro che la legge europea è fatta per evitare di andare in infrazione. Quindi, se vogliamo applicare l'articolo 81 sulla legge europea, non c'è bisogno di discuterne in Parlamento: il sottosegretario Gozi va in sede di Commissione con un commercialista, mette il timbro su tutte le proposte della Commissione europea e non fa perdere soldi e tempo a questo Parlamento per un qualcosa che alla fine ci viene semplicemente negato: discutere nel merito ed eventualmente decidere

L'articolo 1 si compone di due lettere, la lettera *a)* e la lettera *b)*. La lettera *a)* ci impedisce di indicare con un'evidenza cromatica e con una maggior misura delle lettere l'origine dell'olio di oliva. Vorrei allora chiedere a questo Governo per quale motivo il consumatore non dovrebbe scegliere l'olio d'oliva in base all'origine. Questa sarebbe una competizione molto positiva, perché ogni Paese sarebbe spinto a produrre dell'olio di qualità, in modo che un giorno italiano, invece di comprare l'olio italiano, deciderà di comprare l'olio tunisino. Perché no? Si tratta di competizione sulla qualità. Se noi, invece, non consentiamo al consumatore di scegliere in base all'origine dell'olio facciamo uno scippo di democrazia e di libera scelta. La lettera La lettera *b)* è ancora più grave, perché abolisce sull'etichetta la data di scadenza dell'olio d'oliva. d'oliva. Tutte le associazioni ci dicono che l'olio d'oliva, per le sue caratteristiche, deve essere consumato entro diciotto mesi dall'imbottigliamento. In questo caso, invece, la Commissione europea lascia ai produttori la responsabilità della scadenza, senza neanche indicare linee guida. Questo vuol dire che un produttore può decidere può decidere di vendere quell'olio per 150 anni; non solo: questo rimette sul mercato partite di olio scaduto da tempo e quindi abbasserà il prezzo dell'olio e creerà una concorrenza sleale nei confronti dei produttori quindi, ammazza la produzione dell'olio d'oliva di qualità italiano e si inserisce nella linea di azione di questo Governo, che ha consentito l'importazione di olio della Tunisia oltre le quote stabilite, che non è in grado di risolvere l'emergenza xylella in Puglia e che sta facendo di tutto per ammazzare la produzione italiana di olio d'oliva. Questo è solo l'articolo 1.

l'origine del prodotto solo in base allo stabilimento in cui è avvenuta l'ultima trasformazione e ci impedisce di dichiarare l'origine dell'ingrediente primario. Questo significa che se una mozzarella viene prodotta con latte in polvere prodotto in Cina, importato in Tunisia,

timbrati in Italia diventeranno prosciutto cotto *made in Italy*. Se questo vi sembra il *made in Italy*! A me sembra un'emerita schifezza. Non solo è una schifezza dal punto di vista alimentare, è anche una marchetta ai grandi produttori che hanno bisogno di materie prime a basso prezzo, perché devono comunque competere con condizioni di lavoro e di sicurezza alimentare

trasformatori delle aziende italiane, ancora una volta in linea con questo liberismo sfrenato, sancito anche dal TTIP che appoggiate con tanta energia ma che - ci viene detto - sarà, anche questo, un disastro per l'economia italiana. E vi invito tutti alla manifestazione di sabato per dire

coperture che voi andate a trovare aumentando - in maniera anche piuttosto ridicola - l'IVA sui preparati di risotto. Vi prego, un po' di attenzione: questo è un favore sia alle *lobby* dei giochi d'azzardo sia alla criminalità organizzata. La La Commissione europea ci ha richiamato in quanto le vincite conseguite all'estero, anche tramite operatori *on line*, sono soggette alle aliquote progressive dell'IRPEF (parliamo di giochi d'azzardo o comunque di giochi), mentre per quelle conseguite in case di gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, consistente in un prelievo alla fonte nei confronti degli organizzatori dei giochi pari al 10 per State attenti, però: questa è una tassazione sugli organizzatori dei giochi, non su chi vince, quindi la storia della doppia tassazione è un'emerita fesseria. Questo Parlamento aveva due opportunità: o includere nell'IRPEF le vincite sui giochi, anche *on line*, non esteri (sarebbe stata stata la scelta più giusta, perché avrebbe permesso la tracciabilità), oppure espungere dall'IRPEF sia le vincite italiane sia quelle estere. Poiché con questo provvedimento non si tutela chi è affetto da ludopatia e non si tutela la trasparenza, si è fatta la scelta più canaglia: esentare dall'IRPEF anche dal Gruppo M5S)*. Questo è gravissimo, perché nella relazione della Direzione nazionale antimafia presentata in Parlamento - e ricordo che il senatore Mirabelli è membro della Commissione antimafia, eppure ha sostenuto questa schifezza di articolo si legge che «dietro le attività apparentemente legali, come il gioco lecito, si nascondono sempre più fenomeni corruttivi». Sapete perché? Perché la mafia non dà più le mazzette in contanti, piuttosto apre delle case da gioco *on line* e poi paga i suoi addetti tramite vincite fittizie, che questi ultimi non riportano nella dichiarazione dei redditi. Quante volte vi sarà capitato

che in teoria è una persona stimabile, chiederei di fare un ulteriore ragionamento sull'articolo 7, perché è un favore alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, ed un insulto per chi si sta battendo contro la ludopatia. Andiamo avanti, perché queste sono solo alcune delle schifezze. Se è vero che dobbiamo adeguarci all'Unione europea altrimenti andiamo in procedura d'infrazione, non si capisce perché all'articolo 17, adesso diventato articolo 26, andiamo invece in procedura d'infrazione allegramente. La Commissione europea ci aveva chiesto di fissare la data di chiusura della caccia il 20 gennaio anziché il 31 gennaio, per delle specie particolari e protette. facciamo una deroga all'articolo 81, perché tutto sommato dobbiamo proteggere altre *lobby*. Al di là del fatto che abbiamo degli obblighi per l'adempimento alle disposizioni della Commissione europea, è pur vero che voi utilizzate questi obblighi per fare delle emerite schifezze: favorire i grandi distributori, darvi a un liberismo sfrenato per quanto riguarda l'agroalimentare italiano e favorire - perché no - le *lobby* della caccia. A questo punto, vi chiedo di valutare ancora una volta - non l'avete voluto fare in Commissione - il ritiro dell'articolo 1 e dell'articolo 3 che, essendo in fase di preinfrazione, non è necessario recepire in questa sede; vi chiedo di tornare in sede di Commissione europea e trattare ancora per difendere l'agroalimentare italiano

ci ascolterete, almeno una volta, per il bene degli italiani. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la legge europea 2015 si occupa di sanare o evitare le procedure di infrazione. Anche in questo disegno di legge vi è un lungo elenco di disposizioni che riguardano i temi più diversi, che sembrano apparentemente poco importanti (dall'IVA sul basilico, rosmarino e salvia, all'etichettatura del miele, ai preparati per risotti, al prelievo venatorio, di cui abbiamo appena sentito parlare, fino alla tassazione nelle case da gioco, tema altrettanto importante e rilevante) ovvero altri temi di più largo interesse. Tutte tematiche che riguardano la vita dei cittadini e delle aziende, ed è per questa ragione che meritano la nostra attenzione. Come la norma che, all'articolo 1, introduce il disegno di legge che riguarda gli oli d'oliva vergine (di abbiamo appena sentito parlare in Assemblea), che va a penalizzare il *made in Italy*, come sottolineato in questi giorni da tanti esponenti di Forza Italia. Il nostro Paese è, infatti, uno dei maggiori produttori di olio extravergine e i nostri produttori preservano la qualità del prodotto anche attraverso la commercializzazione entro un determinato periodo. È assai singolare che la Commissione ritenga indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della conservazione. Qualunque persona di buon senso sa che una delle regole per preservare le caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva è quella di conservarlo al meglio e per un periodo non troppo lungo. Altro esempio è l'introduzione di regole relative alla etichettatura del miele, che può essere indicato di «produzione della CE», anche se il prodotto è la risultante della miscela di miele di api di differenti Paesi europei, creando così non solo confusione, ma penalizzando il miele *made in Italy*. Sono solo alcuni primi esempi che ci consentono di capire come questa legge europea continui, purtroppo, in modo evidente nel percorso di un'Italia che cerca solo di evitare le procedure di infrazione e le conseguenti sanzioni. È anche la fotografia di un Paese che continua a subire imposizioni dall'Europa e, nel gioco del dare-avere, certamente l'Italia ci rimette non solo in quanto contributore netto, ma addirittura come Paese che, in alcuni casi, è tenuto ad adottare normative più penalizzanti, rispetto all'esistente, per soddisfare le richieste dell'Unione. È il caso di molte delle disposizioni contenute in questa legge europea 2015, che il Senato esamina per primo, a conferma di quella alternanza che vede al momento la legge di delegazione europea all'esame della Camera. Probabilmente va avviata una seria riflessione sullo strumento della legge europea, che pur prevista dalle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, si limita a correggere le norme italiane in conseguenza di procedure già avviate o in fase di avvio in sede europea. Andrebbe fatto, invece, un lavoro a monte per evitare che talune procedure vengano iniziate laddove riguardano, ad esempio, l'inasprimento delle stesse o l'aumento del prelievo fiscale in taluni ambiti (il capo IV, articoli 8-14 del presente disegno di legge, in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato). Un Paese come il nostro, che ha la pressione fiscale tra le più alte d'Europa, dovrebbe almeno evitare di accettare intimazioni che aumentino il livello di imposizione fiscale. Capiamo che in questo momento, in cui il Governo sarà molto probabilmente costretto ad operare una correzione sui conti pubblici, possa fare comodo avere maggiori entrate fiscali. In questo momento, anche quei poco meno di cinque milioni di euro, che sono il gettito stimato dalle modifiche alla aliquota IVA - dal 4 al 10 per cento - applicabile ai preparati per risotti sono importanti. Tra l'altro, la norma scritta dal Governo, prevista dall'articolo 11, sconfessa una disposizione recentissima dell'Agenzia delle entrate del 24 luglio 2014, che confermava l'applicabilità dell'aliquota al 4 Questo modo di operare produce confusione e toglie reddito a molti operatori del settore. Allo stesso modo l'articolo 12 prevede una tassazione su un maggiore imponibile (50 per cento rispetto all'attuale 40) del reddito dei consorzi agrari. Tra l'altro, sono norme che prevedono un'applicazione pregressa al periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e che generano un effetto che si avrà anche sugli utili maturati nell'anno 2015, incidendo giocoforza sui risultati economici dei consorzi dell'anno appena concluso. Queste realtà pagano adesso una penalizzazione che quasi certamente avrà effetti sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti agli agricoltori nei tanti consorzi agrari sparsi in tutta Italia. Vanno poi citate - lo ricordavano alcuni colleghi intervenuti in Assemblea pochi minuti fa - disposizioni come quelle contenute nell'articolo 3, che abrogano l'obbligo di indicazione di effettiva origine dei prodotti sulle confezioni, confondendo in maniera grave i consumatori sul Paese di origine dei prodotti alimentari. È evidente, quindi, che si va a penalizzare ancora una volta l'eccellenza e la specificità della produzione italiana. che l'articolo 21, che riguarda gli aiuti di Stato, introduce una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato. Concludendo, ci sembra che giorno dopo giorno questo nostro Paese stia perdendo sovranità e finisca per adottare una serie di misure pervasive nelle procedure della pubblica amministrazione, oltre che nella vita delle nostre imprese anche in quella dei nostri cittadini. Serve una Italia più autorevole in sede europea, un Paese che non combatta solo per ottenere clausole di flessibilità, che in definitiva vanno a generare nuovo *deficit*, ma un Governo che riesca a difendere quei piccoli e limitati vantaggi, rispetto alle normative europee, che sono la peculiarità, il segreto del successo del *made in Italy* e che, non essendo scritte sulla pietra, possono certamente essere cambiate ed adattate alle nostre esigenze, ma sicuramente non il contrario. È fondamentale, quindi, tutelare l'interesse dell'Italia, salvaguardare il nostro tessuto produttivo, fatto sopratutto di imprese di piccolissime, piccole e medie dimensioni, che producono qualità e fanno eccellenza, molto spesso in nicchie di mercato e che per questo vanno tutelate. Il *made in Italy*, che si è guadagnato fama in tutto il mondo e che l'Europa, al contrario, tende a penalizzare attraverso regole che mortificano la denominazione dei nostri manufatti più tipici, deve essere la bandiera da sventolare e difendere in questa Europa e di cui tutti noi italiani dobbiamo andare fieri.

decisamente più urbani rispetto a quelli oggi espressi da alcuni colleghi. Mi riferisco in particolare alla senatrice Fattori

molto pacata. È stato fatto uno sforzo da parte di tutti per cercare di cogliere anche il punto di vista altrui; infatti, il bello del lavoro nella 14a Commissione, di cui mi onoro di far parte da tre anni, è sempre stato

tutto il provvedimento. Se fossimo in un'aula di tribunale, si sarebbe dovuto dire che era nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Oggi il Senato è stato chiamato a votare senza sapere su cosa stava votando, e trovo che questo sia un fatto assolutamente

Non si è tenuto conto del fatto che esiste uno strumento regolamentare che consente, sia alle Commissioni che all'Assemblea,

5a Commissione si era espressa contrariamente, va detto che anche il suo Gruppo ha votato a favore in quella Commissione, quindi egli oggi ha in qualche modo sfiduciato il suo stesso Gruppo; in ogni caso esistono altri strumenti

a volte, anche lo stupore nei confronti di una politica europea che si preoccupa molto di questioni di dettaglio,

il tipo di Unione europea che vogliamo costruire. È l'Unione europea che abbiamo quando abbandoniamo gli aspetti valoriali e dimentichiamo i valori ispiratori dell'Unione europea. Questo è grave, ma è anche frutto di una politica che si è protratta per almeno dieci anni. L'Unione europea non è una istituzione neutra. Ci sono delle maggioranze, anche politiche. Questo è il frutto, un po' avvelenato, di una Commissione europea dominata da maggioranze di centrodestra e dalla Commissione Barroso, che ha fatto peculiarità dell'Unione europea un aspetto burocratico. Quindi, quando noi oggi lamentiamo, e sentiamo lamentarsi anche altre forze, del fatto che l'Unione europea sia diventata molto burocratica, questa è la logica conseguenza di un certo tipo di politica. Non è un fatto casuale.

violando le norme dei trattati e andando incontro a delle sanzioni che possiamo meglio tutelare l'Unione europea e il nostro Paese. Ha ragione il senatore Tremonti quando invoca il criterio della sussidiarietà.

e si procede, nella cosiddetta fase ascendente, all'attività normativa regolare nelle Commissioni. È lì che noi difendiamo i valori dell'Italia, gli interessi degli italiani e il principio di sussidiarietà. Invocarlo quando siamo nell'ambito della legge europea significa dire una cosa giusta nel posto sbagliato. Quindi, bisognerebbe anche avere il buon senso di scegliere il momento opportuno per fare certe affermazioni anche un po' pirotecniche,

della sedimentazione di una serie di malepolitiche messe in opera non soltanto negli ultimi tre o quattro mesi. Questo è ridicolo perché, in realtà, tutte le infrazioni di cui stiamo parlando risalgono ad anni antecedenti al 2011, quindi ad altre legislature e ad altri Governi. lascia un po' perplessi sentire oggi coloro che erano al Governo quando si sono creati i presupposti per l'infrazione pontificare sul fatto che poi la stessa si è in qualche modo trasformata in una procedura d'infrazione. PD)*. Evitiamo oggi di creare un arretrato ed evitiamo di arrivare sempre all'ultimo momento. È vero che in questa legge europea ci sono delle procedure che non sono ancora arrivate a una procedura di infrazione e che siamo in un caso ancora precedente. Mi domando, però, per quale motivo dovremmo arrivare all'infrazione e per quale motivo dovremmo negoziare sotto la spada di Damocle di una sanzione così consistente. Ieri, nella mia relazione avevo accennato a quali sono le sanzioni, hanno importi assolutamente pesanti. Per ciascuna infrazione l'Italia dovrebbe pagare 8,916 milioni di euro, oltre a una penalità di mora di 10.753 euro al minimo o 645.000 euro al massimo Per quale motivo dovremmo metterci nella condizione di subire questo tipo di penalità e quindi negoziare in ginocchio? Lo domando a coloro che si sono lamentati del fatto che si sia voluta anticipare la procedura. Oggi possiamo trattare a testa alta. Domani negozieremmo negozieremmo in ginocchio. Quindi è assolutamente eccentrica la posizione di chi dice che potevamo ancora aspettare: ma per andare incontro a che cosa? Oggi abbiamo fatto un'azione importante. Abbiamo il *record* storico di riduzione del contenzioso, essendo scesi di quasi 40 40 procedure. Mentre all'inizio del mandato del Governo in carica eravamo a 120 procedure di infrazione, oggi siamo arrivati a 80. Questo è il modo con il quale oggi noi tuteliamo i nostri interessi e quelli degli imprenditori e dei cittadini italiani.

approvato a larga maggioranza un importante ordine del giorno con il quale non soltanto abbiamo dato un'indicazione su come trattare le vincite nelle case da gioco, ma abbiamo anche impegnato il Governo a destinare la tassazione che deriverà dalle vincite del gioco *online* alla cura della ludopatia. Quindi, se c'è una misura che è stata adottata in maniera concreta da parte della Commissione, e quindi del Parlamento, è stata proprio quella di ribadire l'impegno contro la ludopatia,

Signor Presidente, gentili colleghi, sono qui ad illustrare l'ordine del giorno G26.101 a mia firma relativo alla disciplina della sperimentazione animale. L'ordine del giorno è stato presentato in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, facendo tesoro della notizia di giovedì scorso della messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea rispetto al decreto legislativo n. 26 del 2014 con cui abbiamo recepito la direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questa notizia era attesa da quanti tra noi si sono occupati del tema. La scelta della Commissione è un atto dovuto dopo che il Parlamento e il Governo hanno aggiunto limiti alla disciplina, nonostante l'espresso divieto contenuto nella direttiva stessa. Di tutti questi aspetti si è trattato sia nel dibattito pubblico che nelle sedi proprie: penso al parere della Commissione sanità sulla bozza di decreto legislativo del Governo, in cui puntualmente c'è una disamina tecnica e analitica degli aspetti giuridici in contrasto con le norme dell'Unione, parere che richiamo nell'ordine del giorno depositato. Ieri sera, il relatore Cociancich, nell'illustrare il disegno di legge, ci ricordava come dei 38 articoli oggi in discussione ben 16 recano modifiche alla normativa nazionale al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi europei o procedure di infrazione. Il caso della sperimentazione animale appartiene esattamente all'ipotesi presente in questi 16 articoli. Oggi si tratta di prendere atto di questo contenzioso e, se il relatore e il Governo volessero, potrebbero presentare fin da ora un emendamento volto a prevenire ogni procedura di infrazione e soprattutto a mettere i ricercatori italiani in grado di competere ad armi pari con i colleghi europei. Mi rendo però conto che forse operare in questo passaggio parlamentare sia tardi. Pertanto con questo ordine del giorno vorrei impegnare il Governo...

affinché, qualora alla Camera questo disegno di legge venisse modificato, si potesse cogliere l'occasione, fin da questa legge europea, per apportare quelle modifiche legislative che scongiurino la procedura d'infrazione.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono qui per denunciare un fatto: l'altro ieri mattina Mattia Perin, portiere della squadra del Genoa, nonché secondo portiere della nazionale italiana, riaprendo una ferita storica, una delle pagine più buie della storia dell'Italia contemporanea, sul suo profilo di Instagram - lo ha scritto sulla tastiera di una *smartphone*, che forse è l'unica vista nella sua esistenza, fatta tutta di piedi e senza cervello - in occasione di un battibecco con un tifoso del Frosinone - Perin è di Latina e da questo nascono gli sfottò da parte dei dei sostenitori gialloazzurri - ha scritto: «A Vallecorsa cambiò la storia, tuo nonno parla arabo... il mio fondò Littoria!». Il messaggio *shock* fa riferimento alle marocchinate, ovvero agli stupri e alle violenze che subirono non solo le donne, ma l'intera popolazione della provincia di Frosinone da parte delle truppe marocchine inquadrate nel corpo di spedizione francese in Italia. Il paese di Vallecorsa, al quale fa riferimento Perin, fu drammaticamente coinvolto da quegli eventi: ci furono, solo a Vallecorsa, 418 stupri, 29 omicidi e 517 furti. furti. Questa è la storia della marocchinate, quella che ieri ha infamato Perin, un ragazzino viziato. Non importa sapere se quel disgustoso riferimento sia stato fatto per ignoranza o con consapevolezza. È di una gravità inaudita in entrambi i casi. Quella delle marocchinate è una ferita che rimarrà aperta per sempre, e non solo per le popolazioni del basso Lazio. Perin è ignorante in storia e geografia, ignaro anche del fatto che la sua provincia, quella di Latina, ha conosciuto i martiri imposti dai marocchini. Questo episodio non potrà essere archiviato impunemente e non bastano nemmeno le scuse arrivate ieri su Instagram. Non sono sufficienti: il giocatore va sanzionato a livello disciplinare, perché indossa la maglia di quell'Italia, essendo secondo portiere della nazionale italiana, la cui storia ieri ha vergognosamente infangato. Nella competizione sportiva la rivalità fra *club* non deve mai sconfinare: questa volta Perin dimostra una totale insensibilità e una nostalgia assai pericolosa.

Hai toppato, Mattia, e lo hai fatto nel modo più doloroso possibile perché, se con ciò intendevi celebrare la retrocessione del Frosinone, da tifoso del Latina, sappi che hai solo esaltato la tua viltà ed estrema ignoranza di cittadino italiano, quell'Italia che ti pregi di rappresentare, perché sei un bravo portiere, ma che non meriti, in quanto uomo piccolo piccolo. Spero che qualcuno possa avere la bontà di spiegarti quanto accaduto, magari un figlio di quella barbarie o anche un bambino, uno come te, che ha conosciuto la storia dal racconto di un nonno, che magari non ha fondato Littoria, ma che in quei giorni ha sofferto, con l'eco dell'arabo che gli rimbombava nel cervello. *(Applausi

sui 130 dipendenti della società König di Molteno, in provincia di Lecco, si è abbattuto un fulmine a ciel sereno, perché l'ultima proprietà ha deciso senza preavviso di chiudere lo stabilimento. La König è una storica società lecchese, nata nel 1966, che fabbrica e innova nel settore delle catene da neve. Nel 2004 la società è stata acquisita dal gruppo svedese Thule

non è stata preceduta da alcun preavviso né da alcuna comunicazione alle rappresentanze sindacali.

di fronte all'ottimismo sparso a piene mani, a 360 gradi, da parte del *premier* Renzi, quello che si è evidenzia è la cruda realtà. alte tasse e l'alto costo dell'energia incidono sull'alto costo del lavoro e la burocrazia e i lunghi tempi della giustizia amministrativa fanno sì che si moltiplichino i fenomeni di delocalizzazione in tutto il Paese e ormai segnano anche il territorio lecchese che, fino a pochi anni fa, anni fa, non registrava problemi di lavoro e - lo voglio ricordare - la disoccupazione era al 2 per cento. È per questo motivo che ho presentato una interrogazione parlamentare urgente al ministro del lavoro Poletti e al Ministero dello sviluppo economico, ancorché

con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale dove membri e rappresentanti della proprietà e i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, insieme alle istituzioni locali, si incontrino per fronteggiare il problema e addivenire in tempi rapidi a una soluzione positiva di questa annosa vicenda che - ripeto - rischia di lasciare senza lavoro oltre 100 dipendenti del lecchese.

chiedo innanzitutto alla Presidenza di essere autorizzata a lasciare agli atti il documento che ho predisposto che riguarda Human Technopole e che in altre circostanze avrei insistito per leggere. Ho studiato e analizzato l'argomento e ho cercato di capire quali fossero gli aspetti relativi al progetto promosso dal Governo per occupare una parte del *post* Expo con una grande infrastruttura di ricerca, Human Technopole.

E ribadisco in questa sede che l'analisi fatta avrebbe riguardato qualsiasi altro ente prescelto con analoga modalità. In conclusione, vorrei segnalare che ci sono esperienze storiche e analisi politico-economiche che dimostrano che è un errore stabilire per legge quale progetto scientifico sostenere. Le stesse esperienze dimostrano che concentrare il denaro pubblico in poche mani è sbagliato. L'assegnazione continuativa di ingenti somme di denaro pubblico a centri come l'ente beneficiario in questione, che si sottraggono alle rendicontazioni pubbliche e all'amministrazione trasparente, non rispetta l'obbligo etico di fornire prove della ricaduta dell'investimento. Infine, mi permetto di sollevare il fatto che l'ente beneficiario scelto come coordinatore